Grazie,

il termine impedimento ci fa venire in mente il capitolo 2 de «I promessi sposi», il dialogo tra Renzo e don Abbondio che usa il latino per imbrogliarlo, per non celebrare il matrimonio. «Sapete voi quanti siano gl'impedimenti dirimenti?», chiede don Abbondio. «Che vuol ch'io sappia d'impedimenti?», risponde Renzo. «*Error, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, si sis affinis*,... - cominciava don Abbondio, contando sulla punta delle dita.

come don Abbondio. Il vostro *latinorum* è un'espansione senza limiti del legittimo impedimento, e di fronte alle obiezioni tutti - anche il nostro simpatico relatore - rispondete come lui, con un argomento d'autorità o, meglio, con la forza dei numeri. Ma anch'essa, purtroppo per voi, ha dei limiti. Il vostro è un *bluff* come il suo. Alla fine Renzo si sposa e alla fine questo testo incostituzionale cadrà.

«Al fine di garantire il libero e ordinato esercizio delle prerogative e competenze connesse all'esercizio del mandato parlamentare» - quindi, andavamo oltre, per tutti noi parlamentari «ai sensi degli articoli 67 e 68 della Costituzione, la presente legge riconosce priorità assoluta ai procedimenti penali a carico di membri delle Camere, in sede di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi». Il collega Ichino aveva studiato e aveva scritto una bella presentazione di questo emendamento, che ha inserito nel suo sito. Mi limito a citarla (mi aveva fatto l'onore di presentarlo lui, anche se io ero il primo firmatario): «Si otterrà in questo modo il duplice importantissimo risultato di garantire al politico incriminato la possibilità di chiarire immediatamente la propria posizione rendendo conto al Paese del proprio operato e al tempo stesso di evitare che l'ombra dell'accusa si allunghi indebitamente sull'intera durata del suo mandato».

mira a tutelare - come voi fate qui - la separazione dei poteri. Così come il legittimo impedimento è fatto per impedire che il potere giudiziario prevarichi su quello legislativo, è giusto che non ci siano interferenze dal potere legislativo verso quello giudiziario. 1.513 si legge: «Qualora l'avvocato difensore rivesta le funzioni di parlamentare o di titolare di carica di Governo, il Presidente del Consiglio non può avvalersi del legittimo impedimento». Se il Presidente del Consiglio è il primo ad usare un parlamentare per difendersi nel giudiziario, non può poi utilizzare il legittimo impedimento, ossia

perché renderebbe immediatamente operativa la legge, purché ci fosse stata la legge di revisione costituzionale. Si può anche fare prima la legge ordinaria, purché entri in vigore dopo quella costituzionale.

2006 della Corte costituzionale che cosa dice? Ci dice esattamente quanto ha detto il TAR del Lazio, ossia che quando una normativa è incompetente, non è applicabile a quella Regione, ossia non si può applicare. Quindi, non è incostituzionale, non si manda alla Corte perché non si può applicare solo per le Regioni che abbiamo attuato la competenza legislativa. Infatti, il punto 4.4 dei *considerata* in diritto della sentenza "È appena il caso di rilevare, infatti, che l'emanazione di una legge di interpretazione autentica presuppone la sussistenza della potestà legislativa da parte dell'organo legiferante, e che non può ammettersi che tale potestà sopravviva perché «solo l'autore della disposizione che viene interpretata può essere considerato l'unico depositario della volontà legislativa espressa in quella sede»: quella di interpretazione autentica è una legge espressione della potestà legislativa - e non già di una "soggettiva" volontà "chiarificatrice" del suo autore - e pertanto essa, al pari di qualsiasi legge, può provenire soltanto dall'organo attualmente investito di tale potestà, senza che in alcun modo rilevi la qualità di «autore» della legge interpretata". Avendo il Consiglio regionale del Lazio esercitato la competenza, non è più possibile ricorrere all'interpretazione autentica da parte del legislatore statale,

Signora Presidente, il disegno di legge sul legittimo impedimento, che voi questa sera approverete, contiene delle perle di assurdità logica e giuridica, delle perle di vergogna e dei punti di rottura della legittimità costituzionale in modo palese, in maniera manifesta. Per sintesi ripercorro quanto emerso e quanto sarebbe emerso dall'illustrazione dei nostri emendamenti, illustrazione che ci avete impedito con il voto di fiducia. Voi imponete una presunzione assoluta di legittimo impedimento che comporterà un blocco dell'attività giurisdizionale, un allungamento dei tempi processuali, la prevaricazione di un potere - quello Esecutivo - su un altro, quello giurisdizionale. Inoltre, voi create una vera e propria prerogativa, un privilegio per i titolari delle funzioni di governo, prerogativa e privilegio finalizzati a proteggere una singola persona o poche persone dall'esercizio della giurisdizione; privilegio personale creato, inventato mediante una legge ordinaria in spregio assoluto agli articoli 3 e 138 della Costituzione, in spregio soprattutto all'inderogabile principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e davanti al giudice. ulteriore sfregio alla nostra Costituzione per la palese incongruenza e istituzionale irrazionalità di prevedere un privilegio per reati comuni commessi dal *Premier*, sottratti all'esame del giudice, mentre per i reati commessi e giustificati dall'esercizio della funzione di governo tale prerogativa non sussiste. Il tutto è ulteriormente aggravato, dolosamente aggravato dalla piena vostra consapevolezza della necessità di una legge costituzionale, come confessato da voi stessi con l'articolo 2 del disegno di legge. Ma ciò richiederebbe per voi troppo tempo e il popolo italiano boccerebbe con *referendum* questa vostra nefasta iniziativa. Tutto ciò vanificherebbe la necessità - questa sì - per voi assoluta di salvare il Presidente del Consiglio dalle accuse di corruzione e frode. Ma ciò che politicamente e socialmente ci preoccupa di più è il fatto che questo disegno di legge, anziché affrontare i veri problemi del nostro Paese (quelli occupazionali, economici, finanziari, imprenditoriali, infrastrutturali e ambientali), è l'ultima trovata per sollevare il Presidente del Consiglio dalle sue responsabilità penali. La XVI legislatura è iniziata con le vostre norme blocca processi - volevate bloccare circa 100.000 processi - ed è continuata con il lodo Alfano, con le norme sulle intercettazioni telefoniche per bloccare le indagini della polizia e della magistratura, con il disegno di legge sul processo penale contenente norme ancora una volta finalizzate ad ostacolare le indagini di polizia e magistratura e a tutelare il *premier* Berlusconi dalla possibilità che la sentenza di condanna per David Mills sia utilizzata contro lo stesso Berlusconi. Si è continuato con il cosiddetto processo breve, che invece è istituzionalmente lunghissimo, e continuate - e per il momento vi fermate - con il disegno di legge sul legittimo impedimento.

solo parlando - di riforma della giustizia come fa il Ministro della giustizia presente in Aula, quando poi ve ne infischiate letteralmente delle nostre proposte, precise e concrete, forse proprio con l'inconfessabile speranza che il nostro sistema giustizia imploda. imploda. Concludo il mio intervento con una suggestione: quella che avete inserito nel disegno di legge al nostro esame prospettando la necessità di garantire la serenità del Presidente del Consiglio. Provengo da terra veneta, dalla terra della Venezia Serenissima, e serenissimo era il nostro Doge. Forse il presidente Berlusconi ha ambizioni o mire dogali o - peggio ancora - principesche, ma ricordiamoci che serenità non ha mai voluto dire irresponsabilità. Il Doge era serenissimo, ma pienamente responsabile. Invece voi volete un *Premier* irresponsabile, impunito, sottratto ai controlli della legge e della Costituzione. Questa è una manifesta rottura della legalità costituzionale. È la negazione dei principi del nostro Stato democratico. Presidente, colleghi, probabilmente non sarò originale nel mio intervento, ma visto che tutti hanno usato espressioni latine, lo farò anche io: *repetita iuvant*! Pertanto, mi ripeterò su qualche punto a voi molto caro. 22 mesi di provvedimenti per favorire il Presidente del Consiglio, 31 richieste di fiducia, un Parlamento sotto sequestro della maggioranza, sfibrato nelle sue funzioni, espropriato del primario compito legislativo, umiliato per la continua compressione dei tempi di discussione dei provvedimenti.

Ebbene, la protesta dell'Italia dei Valori sarà sempre - ripeto - più ficcante e più estrema perché è l'unico strumento che abbiamo per far sapere le malefatte del Governo e della sua maggioranza. E lo faremo: la pazienza non ci manca e il buon Dio ci assisterà, perché siamo impegnati in una causa buona e giusta. Il Paese è in forte sofferenza. Il Paese - lo abbiamo dimostrato - è nelle condizioni in cui noi plasticamente lo abbiamo rappresentato: con il sedere per terra. Un Paese in difficoltà, corroso dalla corruzione,

Questo è il Paese, e noi siamo impegnati nella difesa soltanto del Presidente del Consiglio e dei suoi Ministri, come al solito più uguali degli altri, dinanzi ad un provvedimento che è, vivaddio, assolutamente incostituzionale. E voi lo sapete bene, perché al vostro interno vi sono giuristi che queste cose le conoscono e le sanno: però bisogna obbedire, perché il principale chiede atti di fede e di obbedienza totale! Questo è un provvedimento vergognoso, e sono ancora più gravi le vergogne e le bugie che il Presidente del Consiglio sta mediaticamente diffondendo, anche in queste ore: un povero perseguitato dalle opposizioni; un povero perseguitato dai giudici; un povero perseguitato, insomma. Egli invece non sa scrivere le leggi, ha consulenti che non lo aiutano a saperle scrivere, vara decreti-legge che non risolvono i problemi suoi e neppure del suo partito: sarebbe bastata una alfabetizzazione dei suoi funzionari di partito e forse le liste sarebbero state presentate in modo trasparente, in modo lineare e sarebbero state accettate senza trucchetti dell'ultima ora, che ogni giorno vengono pubblicati sui giornali e messi in evidenza dalle stesse fonti della maggioranza. L'Italia dei Valori è indignata per questo modo di legiferare, è indignata per questo modo di attentare all'informazione, ormai tutta in ginocchio, perché nessuno sappia, nessuno senta, nessuno veda.

di far conoscere al Paese quello che oggi approvate. Rimarremo, finché sarà possibile rimanere nelle Aule parlamentari con questo clima, ma sappiate, colleghi di maggioranza, sappia la Presidenza, sappiano i colleghi dell'opposizione che non ci fermeremo dinanzi ad ulteriori atti di prevaricazione e di arroganza.

in un Paese normale, per usare un'espressione cara alle opposizioni, non ci sarebbe alcun bisogno di una legge sul legittimo impedimento del *Premier* e dei Ministri. Basterebbe applicare una disposizione contenuta nel nostro codice di rito, l'articolo 420-*ter,* e basterebbe applicare il principio di leale collaborazione tra le istituzioni, tra la magistratura e il Governo, principio che ben avrebbe potuto risolvere tutti i problemi, con la fissazione di un calendario di udienze compatibili con le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, funzioni che ovviamente lo vorrebbero a Palazzo Chigi e non al tribunale di Milano ad esercitare il proprio diritto alla difesa. In un Paese normale, colleghi dell'opposizione,

vi sembra normale un Paese nel quale i due processi penali a carico del *Premier* hanno un calendario di 22 udienze fissate nei prossimi 72 giorni? solo mese di marzo sono state fissate cinque udienze (1° marzo, 8 marzo, 15 marzo, 22 marzo e 29 marzo) nel processo sui diritti televisivi,

Vi sembra normale un Paese nel quale perfino la convocazione del Consiglio dei ministri per approvare un disegno di legge sulla corruzione non assurge a causa di legittimo impedimento

Dobbiamo operare un bilanciamento tra valori ugualmente meritevoli di tutela: l'autonomia della funzione di governo da una parte e l'efficienza della funzione giurisdizionale dall'altra. Tale bilanciamento fra le esigenze del processo penale e quelle della funzionalità delle istituzioni di governo non può che essere operato nel senso che le attività funzionalmente collegate all'esercizio del mandato di governo costituiscano quell'impedimento che legittima non già il sacrificio, ma solo il ritardo della funzione giurisdizionale. In un'operazione così insidiosa come il bilanciamento, che esalta la soggettività e la discrezionalità di chi deve effettuarlo, si ha bisogno di certezze e di oggettività, tanto più nelle ipotesi in cui il bilanciamento pone in causa da una parte la funzione di governo e dall'altra la funzione giurisdizionale. Poiché il bilanciamento, proprio perché connotato da una forte componente discrezionale, ha bisogno di certezze ed oggettività, occorre, in un Paese non normale, che venga effettuato dal legislatore una volta per tutte. In un Paese non normale la certezza del diritto impone di limitare la discrezionalità del giudice nel valutare le cause di assoluto impedimento, identificando un modulo generale di bilanciamento degli interessi in gioco adeguato a tutelare il membro del Governo anche contro l'eventuale esercizio persecutorio della giurisdizione. Ricordo ai colleghi dell'opposizione che il 28 ottobre 1999 l'Ufficio di Presidenza della Camera, sotto l'illuminata presidenza dell'onorevole Violante, deliberò di sollevare un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del giudice di Milano dottor Rossato, che non considerava assoluto impedimento l'esercizio della funzione parlamentare dell'onorevole Previti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 2001 sul caso Previti, ha chiaramente dichiarato che il giudice deve, o meglio dovrebbe, farsi carico delle difficoltà che incontra il titolare di una carica istituzionale a prendere parte a un processo penale, coordinando le esigenze della giustizia con quelle della politica. Ma l'auspicio della Corte in questo Paese non normale è rimasto sulla carta. In questo Paese, se l'impedimento addotto dall'imputato è legato, ad esempio, alle festività religiose, allora va bene. Mi riferisco a un caso realmente verificatosi: un imputato di fede ebraica si è presentato davanti al giudice sostenendo di non poter partecipare al processo perché nel giorno dell'udienza ricorreva una festività religiosa ebraica; in quel caso i giudici hanno riconosciuto il legittimo impedimento per la festività religiosa. Se però l'impedimento addotto è legato agli impegni del *Premier* e alla convocazione del Consiglio dei ministri, allora non va bene per nulla. Allora, in questo Paese non normale, a tipicizzare nell'articolo 1 del disegno di legge in discussione le ipotesi di impedimento connesse alle funzioni di governo il cui espletamento è da ritenersi incompatibile con la possibilità di comparire e di difendersi in giudizio. Si stabilisce in via preventiva ed astratta come il bilanciamento debba essere effettuato per tutti i casi che potranno presentarsi nella realtà. Non si tratta di un'immunità processuale forgiata per il Presidente del Consiglio *(Commenti* *dal Gruppo PD)*: la legge non riguarda le prerogative costituzionali, ma il diritto di difesa del *Premier* ogni volta che lo svolgimento delle sue funzioni ne comprometta la possibilità di partecipare attivamente al processo. Con onestà intellettuale dobbiamo dire che è anche una soluzione ispirata alla filosofia della riduzione del danno, per sottrarre il Governo dagli attacchi di alcuni (per fortuna pochi) giudici. Come ha scritto pochi giorni fa il professor Nicolò Zanon, ordinario di diritto costituzionale a Milano (quindi non un sovversivo), questa legge è «un argine contro la deriva verso la repubblica giudiziaria». Colleghi, un argine va eretto: la politica ha il dovere di erigere questo argine a difesa non solo del prestigio delle istituzioni, delle attribuzioni costituzionali del Governo, ma soprattutto del voto democratico degli elettori che si sono pronunciati due anni fa *(Commenti del circa l'indiscriminata prevalenza delle esigenze della giustizia a detrimento di ogni altro interesse costituzionalmente rilevante appare drastica e forzata. Non ci sono solo i giudici in questo Paese, cari colleghi dell'opposizione: c'è anche il Governo, questa legge tenta, in un Paese non normale, un contemperamento tra l'interesse dello svolgimento della funzione giurisdizionale e l'interesse a governare E trova secondo noi un punto di equilibrio costituzionalmente corretto tra i diversi valori in campo, nella speranza in futuro di un Paese normale, nel quale non ci sia più bisogno di questa legge e nel quale in Parlamento si possa discutere di altro.

Signora Presidente, se il Governo non avesse posto la questione di fiducia, io adesso avrei illustrato i pochi emendamenti presentati e questo mi avrebbe dato modo di esporre esporre al senatore Mazzatorta un'opinione diversa dalla sua. Viceversa, il voto di fiducia mi induce (direi mi costringe) a dare un taglio esclusivamente politico al mio intervento. Dico subito che gli argomenti con i quali ieri sera, in merito all'assenza di Berlusconi, il senatore Quagliariello ha risposto alla senatrice Finocchiaro non mi hanno convinto. Lo dico adesso al senatore Gasparri, perché il senatore Quagliariello non è in Aula: in questa legislatura il presidente Berlusconi non ha partecipato a nessun dibattito in Senato, mentre ha trovato molto tempo per fare cose per lui certamente più gradevoli. Pertanto, la questione è quella della totale assenza di Berlusconi dai lavori parlamentari e ciò, assieme al trasferimento della sede del Governo da Palazzo Chigi a casa sua, la dice lunga su quale sia il senso dello Stato del nostro Presidente del Consiglio. Archiviato questo argomento, possiamo dire che in nessun Paese democratico accade quello che sta accadendo adesso in Italia. So bene che nessun argomento, nemmeno il migliore, può convincere i senatori della maggioranza a votare contro un provvedimento incostituzionale che serve a liberare Berlusconi da un contenzioso giudiziario che dura da più di 40 anni. Sottolineo che dura da più di 40 anni per ricordare che Berlusconi non è vittima di una persecuzione giudiziaria in quanto uomo politico,

escluso il senatore Mazzatorta, mi sembra che non vi siano stati molti altri della maggioranza iscritti a parlare. Se per una misura di questa importanza la maggioranza non presenta emendamenti e parla così poco in Aula vuol dire che c'è un ordine

approvare il provvedimento nell'esatta stesura con cui lo ha approvato la Camera. Debbo dire che per me la decisione di porre la fiducia non è stata una sorpresa, perché negli ultimi tempi l'ansia di Berlusconi è diventata molto evidente. Credo che ne avremo molte manifestazioni nel prossimo futuro,

il modo con cui la maggioranza sforna continuamente leggi e leggine per proteggere il suo *leader*, ma ancora prima denunciamo le condizioni nelle quali Berlusconi sta riducendo lo Stato italiano: questa è la vera denuncia che dobbiamo fare in Senato. Debbo dirvi che sono preoccupato di questo ed ho paura per questo: ho paura perché vedo la gravità delle conseguenze sul nostro Paese di un quindicennio nel quale Berlusconi o ha governato o ha impedito che altri governassero.

e che siamo andati ormai molto al di là dello scandalo endemico del suo conflitto di interessi e molto al di là dei rischi per la nostra stessa sicurezza derivanti dai suoi eccessi personali. Emerge ormai sempre più evidente il pericolo più grave che è rappresentato - appunto - dallo sgretolamento dello Stato. Il provvedimento incostituzionale sul legittimo impedimento è solo l'ultimo tassello di questo processo di sradicamento dell'idea dell'idea di legalità. Questa mattina il senatore D'Ambrosio in un intervento veramente bello, per il quale mi voglio complimentare con lui, ha ricordato che il provvedimento sul legittimo impedimento arriva dopo le leggi sulle rogatorie internazionali, sul falso in bilancio e sul legittimo sospetto. Aggiungo che esso arriva anche dopo le leggi sul condono fiscale, dopo il decreto per salvare Retequattro e dopo la legge Gasparri, dopo la riduzione dei termini di prescrizione di cui ha recentemente beneficiato l'avvocato Mills, Mills, dopo il disegno di legge sul processo breve, dopo il lodo Schifani e, infine, dopo il lodo Alfano. Questo spappolamento dello Stato non si ferma però a questo ambito di distruzione della legalità, perché ad esso contribuisce anche quel mix micidiale ed abbondante di decreti-legge, maxiemendamenti e voti di fiducia che sta letteralmente capovolgendo il rapporto tra Governo e Parlamento, nonché lo stravolgimento delle fonti di diritto, con l'abuso delle ordinanze di protezione civile, che hanno forza di legge fuori da ogni emergenza. Vi contribuisce, ancora, lo sprezzo del Presidente del Consiglio nei confronti delle autorità costituzionali di garanzia soltanto le dichiarazioni di Berlusconi a Bonn contro il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale) oltre allo sprezzo contro singoli magistrati e contro la magistratura intera, che è stata definita «banda talebana». contribuisce altresì l'abuso dello *spoils system* politico negli uffici dello Stato, nelle aziende pubbliche e nella televisione pubblica, che determina quella che Giuliano Ferrara ha brillantemente definito «degenerazione cortigiana». Lo ha detto Giuliano Ferrara, non lo sto dicendo io. Stato la trasformazione in società per azioni di pezzi importanti dello Stato stesso, nonché la sempre più profonda spaccatura tra Nord e Sud indotta dalle politiche della Lega e del Governo, che mette a rischio l'unità nazionale. contribuisce poi la legge elettorale del 2005, che riduce drasticamente le scelte degli elettori ed infine, adesso, il decreto-legge emanato per salvare la lista irregolare del PdL nel Lazio, un decreto che lo stesso TAR del Lazio

mi auguro che assista a questo intervento tramite circuito chiuso del Senato - ricorderei al Presidente del Senato che pochi giorni fa, fa, avendo ben presenti le irregolarità elettorali del suo partito, si augurava che la sostanza potesse prevalere sulla forma comunicava al Paese di acconsentire ad una politica governativa fatta di leggi, sanatorie *ex post* che, invece, come Presidente del Senato ha il dovere di combattere. combattere. Questa storia del rapporto tra forma e sostanza è molto strana perché il presidente Schifani ha sostenuto la sostanza contro la forma finché non è stato emanato un decreto-legge pro lista PdL. Naturalmente, adesso che il decreto-legge è stato emanato immagino che dovrà sostenere la forma contro la sostanza, la forma del decreto contro la sostanza delle irregolarità elettorali. IdV)*. Nella speranza che il presidente Schifani mi ascolti, voglio dirgli - e glielo voglio dire in modo leale - che io ho tutto l'interesse politico e anche la volontà personale di tenerlo fuori dalla polemica politica. Ma deve darmi la possibilità di tenerlo fuori della polemica politica dimostrando di saper difendere i diritti dell'opposizione, almeno nella stessa misura e con la stessa tenacia con le quali sostiene le esigenze del Governo. Mi sono meravigliato che, secondo l'ultima moda, anche questo disegno di legge sul legittimo impedimento non sia stato definito una norma interpretativa. Berlusconi ci ha abituato al disprezzo delle regole, ma anche a un modo tartufesco di camuffare la realtà, di mascherarla, calunniando gli avversari e lodando se stesso. E la trovata di deformare l'ordinamento, sostenendo che lo si sta soltanto interpretando, la trovo davvero stupefacente al massimo grado. Termino il mio intervento ricordando gli equivoci dei rapporti internazionali del presidente Berlusconi. Negli ultimi mesi lo abbiamo visto occupato in una singolare visita di Stato del colonnello Gheddafi, soggiornare una settimana nella dacia di Putin per trattare questioni su cui ancora non è venuto in Parlamento a riferire. Ha fatto una visita apparentemente improvvisa in Bielorussia, dove Lukashenko gli avrebbe consegnato incartamenti di cui il Parlamento non ha avuto finora notizia. È andato improvvisamente - non lo aspettavano - in Turchia, dove si è occupato di gasdotti, in assoluto scollegamento dalle politiche energetiche dell'Unione europea che, al contrario di Berlusconi, è molto preoccupata dell'eccessiva dipendenza energetica da un'unica fonte, la Russia, e che di conseguenza ci chiede di diversificare. Ce n'è abbastanza perché il Senato si chieda se questi siano atti della nostra politica estera, della politica estera dell'Italia, o siano iniziative personali dell'onorevole Berlusconi. Noi sappiamo che quando Berlusconi andrà via - perché andrà via ad un certo momento - lascerà uno Stato scardinato nelle sue funzioni più rilevanti. rilevanti. Mi rivolgo allora ai senatori della maggioranza, a quelli presenti. Tra poco, votando la fiducia non approverete soltanto la legge incostituzionale sul legittimo impedimento: voi esprimerete la fiducia a questo insieme di politiche del Governo e vi assumerete con questo voto la vostra parte di responsabilità negli effetti distruttivi di queste politiche. Ricordo modestamente, ma sinceramente che non può esserci nessuna esigenza politica, come non ci può essere nessun *leader*, nemmeno il più potente, le cui vicende personali possano giustificare l'approvazione da parte del Parlamento di misure i cui effetti sfascino lo Stato e distruggano la Repubblica. Per noi in Parlamento l'onore politico è tutto, e io vi chiedo di non rinunciare a cuor leggero all'onore politico. *(Vivi,

e lascio terminare questi applausi che, ovviamente, sono doverosi per quanto riguarda la posizione politica dei nostri contraddittori. Avrei avuto piacere che fosse presente il senatore Ceccanti, perché da professore di diritto costituzionale già gli imputai di essere diventato professore di statistica; oggi è diventato professore di letteratura,

specificazioni applicate a situazioni delicate e forti come quella della quale stiamo discutendo. nonostante il ricorso intellettuale a Manzoni e ai Promessi Sposi e a quelle che furono evidenziate come esercitazioni di brocardi da parte di Azzeccagarbugli, difficilmente si arriva alla materia del contendere politico.

nei grandi termini della Provvidenza. Abbiamo bisogno noi di concetti così elevati quando andiamo a discutere di un provvedimento come questo, in materia di legittimo impedimento? Credo di no, ma forse sì. Quando certe leggi diventano in qualche modo oggetto di un giudizio di Dio va tutto bene, ma bisogna ovviamente rispettare i diversi punti di vista.

Vi sono poi situazioni culturali intermedie. Ieri ho avuto modo di comprare l'ultimissimo libro di Travaglio,

ad oggi, critiche incredibili sulla politica italiana, che non fanno sconti né al centrodestra, né al centrosinistra. Se ci si mette nella posizione di Travaglio, niente è andato bene, niente è stato etico, tutto è stato portato verso posizioni forti ed interessi di parte. Mi piacerebbe che Travaglio diventasse Presidente del Consiglio perché vedremmo come riuscirebbe a risolvere i problemi di uno Stato. Ma, come sappiamo, ed è inutile dirlo, uno un'entità estremamente complessa, che deve curarsi di enormi interessi, che deve mediare, che deve andare avanti, che deve riuscire a contrastare situazioni di tutti i tipi. Allora, il giustizialismo puro, la critica totale non ha senso. Quando qualcuno, un uomo che stimo molto come il senatore Zanda, attacca persino il presidente Schifani, in qualche modo travalica la sua posizione di Vice Capogruppo di un importante partito. Il presidente Schifani fa tutto il possibile per conservare in quest'Aula la garanzia dell'imparzialità ci riesce a mio parere al 100 per cento; se poi c'è qualche momento in cui l'opposizione non è d'accordo, fa parte della fisiologia del reggimento da Presidente di una Assemblea così complessa. Quindi, al presidente Schifani va tutta la nostra stima e sono convinto che, sotto sotto, al di là della retorica degli interventi di contrasto, anche voi la pensate come me. Berlusconi certamente è la vostra bestia nera, perché ha introdotto in questo Paese delle novità che non sarebbero piaciute ad Occhetto e continuano a non piacere al centrosinistra. Occhetto aveva attivato la sua "gioiosa macchina da guerra" sicuro di vincere: Berlusconi è sceso in campo e in tre mesi ha cambiato questo Paese, e - a nostro avviso - lo ha cambiato in meglio! Tutto quello che accade negli anni dobbiamo imputarlo a questa diversissima posizione politica. Noi riteniamo che il centrosinistra sia l'espressione del conservatorismo e che la nostra parte politica sia invece tesa alla novità, all'innovazione e ad una garbata risoluzione. Lo dirà la storia chi ha ragione, non possiamo dircelo fra noi. È chiaro che voi avete tutta una serie di posizioni di contrasto alle nostre, e meno male: se non ci fossero forti posizioni di contrasto vorrebbe dire che c'è una massa indefinita e grigia nella politica, che a noi non piacerebbe. Vogliamo metterci di fronte all'opposizione in termini che per noi sono fortemente costruttivi e fortemente innovatori. Capisco che queste parole non possono piacervi, ma mi auguro che siano del tutto condivise dai colleghi parlamentari che mi sono intorno. Stiamo giocando da anni una partita politica nella quale riteniamo di poter cambiare il Paese e di averlo in parte cambiato. Voi invece pensate che tutto quello che facciamo sia in qualche modo interessato, soprattutto con riguardo a Berlusconi. Non è vero! Abbiamo visto il Presidente del Consiglio raggiunto da una comunicazione giudiziaria, dopo qualche mese dalla vittoria nelle elezioni del 1994, in anticipo sul «Corriere della Sera», e abbiamo capito che non stava bene a troppi la novità della nostra vittoria e delle nostre logiche di cambiamento.

persino serio da parte del centrosinistra, perché non vedo aperture intellettuali significative. Non vedo nessuno che in qualche modo si ponga il problema chiedendosi: avrà ragione Berlusconi? Avranno ragione i berlusconiani? Io vi dico che noi siamo talmente convinti della nostra posizione politica, che ormai da quindici anni sosteniamo tutta una serie di logiche non perché ci danno degli ordini, come qualcuno ha detto... BOSCETTO *(PdL)*. Non ci sarebbe motivo, non ci sarebbe nessuna nostra posizione di lucro attivo. Noi sosteniamo questa politica perché siamo convinti che sia la politica giusta. Accolgo questi applausi ironici,

lungo tempo ormai ci segue e avete timore di quello che accadrà alle prossime elezioni regionali, che avete cercato in tutti i modi di

regionali. Avremo poi davanti a noi tre anni: in quel momento si capirà cosa si può fare in questo Paese per migliorarlo dalle fondamenta. E lì allora voi dovrete partecipare alle grandi riforme riguardanti questo Paese. Vedremo se lo farete. Vedremo se, dopo questi due anni di schermaglie recenti, ci sarà la volontà di soffermarsi a migliorare il Paese. Poi nel 2013 vinca chi vinca; ma sulla base di un lavoro serio fatto da tutti. Pensare e dire, com'è stato detto, che Berlusconi ha scardinato e sta scardinando il Paese è un semplice artifizio retorico. Noi riteniamo che questo Paese, anche attraverso le ultime esperienze, sia stato retto con mano salda dal Governo Berlusconi. Noi abbiamo risolto e stiamo risolvendo problemi forti, soprattutto in economia, che non so come avrebbe potuto risolvere un vostro Governo, che ha dato purtroppo una pessima prova di sé, con tutta la stima per Prodi, nei 18 mesi mesi trascorsi dal 2006 al 2008. Voi non riuscivate ad approvare provvedimenti indispensabili (mi viene in mente un certo decreto sicurezza) perché le divisioni al vostro interno non permettevano di realizzare nulla. Il Paese questa vostra esperienza governativa l'ha vissuta, e non vuole ripeterla. Quando, dopo aver approvato questo provvedimento sul legittimo impedimento alla Camera, voi presentate al Senato 1.500 emendamenti, date evidentemente la prova di non voler discutere: su quei dieci emendamenti fondamentali, sui quali pure si sarebbe potuto discutere: date la prova palese di un ostruzionismo direi addirittura fine a se stesso, perché 1.500 emendamenti sono la prova provata

capisce poco quello che succede nelle Aule parlamentari. Ed è grave questo aspetto: non siamo mai riusciti, in tanti anni, a far capire al Paese come lavorano seriamente i parlamentari seri.

Qui, se non si avessero i decreti-legge, le leggi di conversione ed anche - se è il caso - le ordinanze di protezione civile, non si riuscirebbe in alcun modo a stare dietro alla vita quotidiana del Paese. Il Paese ha bisogno di velocità, mentre abbiamo regolamenti che non sono in grado di consentirla. Se avessimo dovuto votare 1.500 emendamenti nell'Aula del Senato, avremmo passato giornate a discuterli, salvo ghigliottine che,

qui ci saremmo ingaglioffiti, uno dopo l'altro, su una serie di emendamenti, molti dei quali sono stati decisamente creati dagli uffici legislativi che, con la tecnica del canguro, riescono a costruirne a iosa per poi vederseli eventualmente eliminati

duca né in quelli così belli che pure alla fine servono poco alla conclusione dei nostri lavori.

ha posto la questione di fiducia. Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

Palma,

Rossi Nicola, Rossi Paolo,

Non lo ripeto,

Spadoni Urbani, Speziali, Stancanelli,

sciupata, un'occasione che poteva aiutarci a venir fuori dalle secche di una continua, logorante ed innaturale lotta muscolare, che tiene il Paese ostaggio di divisioni cercate in maniera troppo sistematica per non rivestire una qualche funzione strategica. La verità è che questo bipolarismo si regge e si alimenta sul continuo scontro, sulle piazzate, sulle esasperazioni ed il fatto che queste divisioni rappresentino un problema insormontabile per affrontare per affrontare e provare a risolvere le tante questioni che piegano e soffocano le migliori energie della nostra società, ormai non sembra interessare più nessuno. Ancora una volta, quello che per condizioni date poteva essere un terreno praticabile per ricercare una prova di dialogo e di confronto parlamentare, si è trasformato in un esercizio di arroganza della maggioranza; eppure le condizioni c'erano tutte. Nonostante il provvedimento presenti evidenti forzature e non si scorgano affatto ragioni di interesse generale - anzi, se mai si evidenziano forti contraddizioni rispetto ai principi di uguaglianza e di giustizia nonostante tutto ciò, c'era una disponibilità evidente di parte dell'opposizione ad affrontare il provvedimento, magari utilizzando l'approccio, per così dire, del minor danno possibile. Del resto è ormai evidente come in Italia le vicende giudiziarie personali del Capo del Governo rischiano di compromettere definitivamente l'ordinamento generale. L'Italia ha scelto una maggioranza e un *leader* di Governo che, a differenza di tutti gli altri cittadini, non vuole mettere piede nelle aule dei tribunali per difendersi nei processi che lo riguardano: si ritiene in qualche modo legittimato in questo comportamento dal consenso popolare che, in modo assolutamente opinabile, riesce a tradurre persino in una sorta di diritto all'impunità. È con questa impostazione che ormai da anni, e con più provvedimenti, si stanno modificando in peggio norme generali, tenendo bloccate a confrontarsi sulle esigenze e sulla serenità individuale del *Premier*

sarà anche la riforma dell'immunità, ma molto dipenderà dalla fervida immaginazione dei consiglieri giuridici del *Premier*, presenti in massa nelle aule parlamentari. Ma perché non si è voluto cogliere - magari anche strumentalmente - una sostanziale differenza esistente tra le posizioni delle opposizioni sull'argomento? È noto che non tutta l'opposizione è schierata con atteggiamenti di pregiudiziale ostilità antiberlusconiana o su posizioni radicali e giustizialiste. Ed allora perché si è tentato di accreditare ancora una volta le posizioni più ruvide e più spigolose, più inconciliabili? Forse perché queste contrapposizioni non servono solo al *Premier* e alla risoluzione delle sue personali vicende giudiziarie, ma anche ad alimentare, in particolare alla vigilia di una campagna elettorale regionale particolarmente delicata, un sorta di bipolarismo sterile che in questi anni di applicazione italiana ha fatto retrocedere e non avanzare l'intero Paese. Del resto, la parte dell'opposizione più dialogante chiedeva solo di evitare inutili forzature, che lasciassero uno sfregio permanente al nostro ordinamento. Chiedeva di risolvere il problema con giudizio e con il senso del limite e delle proporzioni, affrontandolo insieme nelle sedi parlamentari Ed invece la domanda su fin dove la collettività può correre dei rischi affinché sia garantita la tutela della serenità del Presidente del Consiglio e dei Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, è stata soffocata e annullata dalla ennesima fiducia che apre altre ferite, provoca altre lacerazioni, rende impossibile lo stesso confronto. È stato già spiegato che siamo davanti ad un provvedimento che verrà sicuramente dichiarato incostituzionale. Non lo ripeto, troppi lo hanno ripetuto in discussione generale. Tutto questo lo sa bene il Governo, lo sa bene il Guardasigilli che è corso a spiegarci che le leggi le fa il Parlamento; lo sappiamo, ma sappiamo bene il limite costituzionale di questo provvedimento. È evidente che si confida sui tempi lunghi del pronunciamento di incostituzionalità. Si produce una legge con la consapevolezza che si tratta di un provvedimento illegittimo che verrà annullato. Ma può il legislatore dare questo esempio al Paese? Non siamo di fronte ad un evidente e chiaro abuso del proprio potere? Che cosa è diventato questo ramo del Parlamento, costretto a votare la fiducia su un atto palesemente illegittimo che violenta, mortifica, dissacra la stessa funzione legislativa dei senatori? Quando le leggi sono così palesemente anticostituzionali ed illegittime esiste un diritto e un dovere a contestarle. Con tutti i mezzi quelli leciti, quelli possibili e quelli corretti. Di fatto il messaggio che arriva al Paese è devastante. Con i nostri cittadini alle prese con i mille problemi quotidiani, che la crisi ha amplificato, noi continuiamo a tenere il Parlamento impegnato a discutere per l'ennesima volta dei problemi giudiziari personali suoi nella consapevolezza, Presidente, che nemmeno questa volta sarà l'ultima volta. Ormai il grado di sopportazione che si registra nel Paese ha superato il livello di guardia ed anche i vostri sondaggi stanno là a dimostrarlo. Molti episodi, compresi gli ultimi scandali, hanno finito per aumentare il discredito nei confronti della politica e delle istituzioni. Per favore, colleghi della maggioranza, finitela di abusare della pazienza dei nostri concittadini. Il Paese conserva ancora le energie necessarie per affrontare con serenità il futuro. Ma non esiste democrazia, non esiste coesione sociale o convivenza possibile senza un reale rispetto per gli equilibri tra i diversi poteri chiamati a convivere e che devono convergere su obiettivi comuni. Quegli equilibri, nel nostro Paese esistono, sono stati costruiti faticosamente in anni ed anni di gesti generosi e rispettosi dell'interesse generale. Continuare a produrre strappi, lacerazioni forzature rischia di far saltare tutto. Ed è per queste ragioni, per le nostre ragioni, legate esclusivamente all'interesse generale e collettivo del Paese, e non per cieco pregiudizio antiberlusconiano che, come Alleanza per l'Italia, non abbiamo condiviso questo provvedimento e continueremo a manifestare in ogni sede il nostro dissenso nel merito.

come peraltro in precedenza aveva già fatto con il cosiddetto lodo Schifani sulla sospensione dei processi a carico delle alte cariche dello Stato. Da quel momento l'agenda politica è stata dettata dalle discussioni in materia di giustizia, con la presentazione o la velocizzazione nel calendario dei lavori parlamentari di una serie di proposte per molti aspetti criticabili, come la riforma delle intercettazioni, il processo breve, gli interventi sulla funzionalità del sistema giudiziario, la riforma del processo penale. Questo modo di fare, cari colleghi (interventi immediati, piegati alle individuali esigenze del *Premier*, non ragionati e non condivisi in una materia nella quale la condivisione delle scelte e la discussione deve essere fondamentale) ha in sé un'altissima probabilità di cagionare danni rilevanti al nostro sistema giudiziario e di affossarlo definitivamente, mentre, al contrario, esso meriterebbe un ampio e illuminato intervento riformatore. Per impedire la prosecuzione di quest'attività demolitrice del sistema, l'Unione di Centro si era fatta promotrice alla Camera dei deputati di un'iniziativa, per così dire, di pacificazione, ossia di una norma che regolasse temporaneamente, per il tempo necessario ad aggiornare le regole costituzionali in materia, il rapporto tra il Presidente del Consiglio e la magistratura. Questa è infatti la vera causa che ha bloccato l'attività parlamentare e l'intera azione di Governo nelle secche della questione giustizia, utilizzata spesso senza reale volontà di miglioramento del sistema ma come grimaldello per coprire ogni sorta di nefandezza. Come ebbe ad affermare il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, scrivendo nel 2008 al CSM e alla magistratura, è intercorsa una stagione in cui il potere giudiziario ha talora invaso l'autonomia della politica e viceversa; è forse giunto il momento di iniziare una nuova stagione, quella appunto dell'equilibrio. Noi siamo grati al Capo dello Stato per il difficile lavoro che è chiamato a fare e siamo a lui grati sempre, indipendentemente dal vantaggio politico che le sue decisioni possano determinare. *(Applausi dai Gruppi che deve mostrare maggior rispetto nei confronti di Giorgio Napolitano, perché ha sempre guidato - sempre guidato - con equilibrio le nostre istituzioni repubblicane, spesse volte martellate dalla insensatezza e dalla insensibilità giuridica e istituzionale di troppi. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-IS-Aut e PD)*. Lo vogliamo dire all'Italia dei Valori, che spesso ha mostrato e mostra irresponsabile disprezzo per la funzione di garante dell'unità nazionale che il Presidente della Repubblica svolge. Per la verità, la cultura giuridica dell'Italia dei Valori è speculare a quella del Popolo della Libertà, sono due facce populiste e antigiuridiche della stessa medaglia. L'Italia ha bisogno di meglio, di equilibrio e di efficiente moderazione. Un equilibrio che non può trasformarsi in equilibrismo e non può più fondarsi, ovviamente, sul recupero dell'istituto dell'immunità parlamentare, ma che può, nel solco dell'insegnamento e delle indicazioni che provengono dalla Corte costituzionale, essere fondato anche su sistemi di tutela temporanea e funzionale dell'attività di governo e di alta amministrazione del Presidente del Consiglio.

del Presidente del Consiglio dei ministri; una proposta tecnicamente corretta e che non fosse oggetto di abusive estensioni. In realtà, e come al solito, cari colleghi della maggioranza, vi siete allargati, abusando della disponibilità di una parte dell'opposizione che pensa che il conflitto tra politica e magistratura debba essere superato e non utilizzato come una clava in danno del Paese. Noi volevamo una norma che consentisse solo al *Premier* di anteporre temporaneamente alle esigenze della giustizia quelle del Paese e voi la avete estesa ai Ministri; e volevate pure, secondo la nota locuzione latina *melius* *abundare* *quam deficere*, estenderla ai Vice Ministri ed ai Sottosegretari. Noi volevamo che il legittimo impedimento, come causa eccezionale di rinvio dei processi, fosse circoscritto obiettivamente ai casi in cui il Presidente del Consiglio è chiamato a svolgere le funzioni che la Costituzione e la legge gli impongono; voi invece lo avete esteso così tanto che basta un'autocertificazione dell'onorevole Berlusconi per rinviare l'udienza per sei mesi e considerare coessenziale alle funzioni presidenziali anche la partecipazione del Capo dell'Esecutivo ad una partita del Milan o a una festa a Palazzo Grazioli. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Un provvedimento così non ci piaceva e non ci piace; e non è il nostro, caro collega Quagliariello. Nonostante ciò, abbiamo presentato pochi emendamenti, sette, per ricondurlo alla sua giusta ed accettabile formulazione. La risposta del Governo è stata la questione di fiducia, che ha reso impossibile il confronto parlamentare e quindi la discussione delle nostre proposte. Cari colleghi della maggioranza, voi avete chiuso il dialogo e il confronto. E non è certo l'eccesso di zelo nella fase emendativa, diciamo così, degli altri Gruppi di opposizione ad avervi costretto a sbatterci la porta in faccia, ma l'urgenza di incassare questo modesto risultato e di rifugiarvi in piazza, aumentando il livello dello scontro politico per far dimenticare, soprattutto ai vostri elettori, i clamorosi errori di cui siete responsabili e le drammatiche inefficienze di questi due anni di Governo. Essendo piccolo, come dice la collega Finocchiaro, lungi da me l'idea di difendere i colleghi del Partito Democratico, ma non penso che a loro possa essere imputato di aver fatto ostruzionismo o una vera "opposizione" su questo provvedimento (anche se qualche iniziativa può dare spazio ad alibi della maggioranza), perché, se fosse stato così, avremmo avuto un altro calendario dei lavori. Né potete scambiare per ostruzionismo la presentazione di emendamenti fotocopia, facilmente eliminabili con i poteri che il Regolamento conferisce al Presidente del Senato. In realtà, nessuno ha pensato pretestuosamente di mettervi i bastoni tra le ruote; certamente non noi e devo dire neanche il PD, anche perché siete sempre bravi ed insuperabili a farlo da soli. Il problema reale è che la fiducia da voi imposta segna un cambio di passo e di atteggiamento nella discussione sulla giustizia. Avete abbandonato la strada del dialogo e del confronto con le opposizioni, per prendere la solita e dannosa scorciatoia, quella della piazza. La stessa piazza cui impropriamente hanno fatto e continuano a fare ricorso altri Gruppi di opposizione. Per carità: massimo rispetto e considerazione per i cittadini che protestano e che manifestano liberamente ‑ grazie a Dio ‑ il loro pensiero, ma la politica ha altro tipo di responsabilità, sia quella di maggioranza che quella di opposizione. Non può esaurire la propria azione politica, di governo o di opposizione, buttandola sempre in caciara e sequestrando il Paese in un'interminabile rissa su tutto, perché nulla cambi. Noi tutti abbiamo il dovere di dare risposte nelle istituzioni e per conto delle istituzioni che rappresentiamo. Il ricorso alla piazza è sbagliato, cari colleghi dell'opposizione, perché è qui in Parlamento che dobbiamo avere la capacità di far emergere, con le nostre proposte, le evidenti ed irreversibili contraddizioni della maggioranza. L'idea di accedere alla tesi del legittimo impedimento nella sua versione casta e pura (diciamo così), se da voi condivisa, avrebbe separato definitivamente il destino del Presidente del Consiglio da quello della sua corte, una parte della quale è obiettivamente indifendibile. Avrebbe consentito di far cadere l'alibi dell'accanimento giudiziario nei confronti del Capo dell'Esecutivo - che c'è stato e c'è - come discriminante della dialettica tra maggioranza ed opposizione, spingendo l'onorevole Berlusconi a confrontarsi sulle cose fatte e, soprattutto, sulle cose non fatte, ad esempio sulla profonda crisi economica del nostro Paese (la più grave dal dopoguerra ad oggi), sulla crescita esponenziale della disoccupazione e sul costante logoramento del nostro sistema produttivo. Il ricorso alla piazza, signori della maggioranza e del Governo, è la più evidente tra le dichiarazioni di fallimento della vostra azione politica dentro le istituzioni. State sbagliando e continuate a farlo,

(gestite con ignoranza, improvvisazione, spocchia e prepotenza), dimostra tutta la debolezza della vostra maggioranza ed un lento ma costante processo di logoramento della *leadership* dell'onorevole Berlusconi. Questo modo di fare ci costringe ad assistere attoniti, ad esempio, allo spettacolo indecoroso che induce ormai ogni rubagalline preso con le mani nel sacco a dichiararsi prigioniero politico e perseguitato dai giudici; allo spettacolo che rende l'ultimo luogotenente del regno vittima della persecuzione giudiziaria, anziché destinatario di pedate nel sedere da parte dei suoi capi, con tanto di scuse agli elettori, quando non sa presentare le liste per tempo e non rispetta le regole. A proposito, che fine ha fatto il pacchetto anticorruzione del Governo? Mi sembra che al riguardo il Consiglio dei ministri abbia deliberato solo un comunicato stampa. Non è un bello spettacolo quello che ci state proponendo, colleghi della maggioranza. Esso ci rappresenta un Capo dell'Esecutivo debole e prigioniero dei suoi cortigiani (non tutti al di sopra di ogni sospetto), incapace di parlare il linguaggio della verità, ma costretto dagli eventi e dai disastri provocati dalla sua allegra brigata ad attaccare gli altri e trovare sempre un capro espiatorio su cui scaricare la colpa delle cose non fatte. un Capo dell'Esecutivo vittima dei suoi cavilli legali. Ho personale simpatia per il senatore Longo e per l'onorevole Ghedini, ma proprio per restare alla mia giovane - anche se non più tenera - età, mi sembrano tanto il mago Gargamella e la sua gatta Birba, che tentano di catturare i Puffi con ogni forma di espediente e di trucco, fallendo sempre miseramente. La loro pregevole arte forense, unita alla spocchia e alla prepotenza della maggioranza del gruppo dirigente del Popolo della Libertà, ha reso il Presidente del Consiglio simile al personaggio di Wile E. Coyote, vittima del suo ingegno, che gli procura però, il più delle volte, soltanto un volo nella gola di un *canyon*. Non potete continuare su questa strada, perché arrecate danno al Paese a causa del vostro non governo: con il voto di fiducia ci avete messo di fronte alla logica devastante del prendere o lasciare, ma questo ennesimo errore politico e legislativo ve lo lasciamo volentieri ed esprimiamo quindi voto

il Presidente della Repubblica ha ricordato, appena due giorni fa, che esiste uno straordinario complesso di valori e principi condiviso dal popolo e racchiuso nella nostra Costituzione. C'è però una linea di discrimine tra chi condivide tale complesso di valori e principi e chi invece è insofferente ad esso: si avverte, infatti, il segno profondo dello sfarinamento della legge e dello sgretolamento dell'architettura del nostro Stato. La legge, da espressione applicata della democrazia, viene retrocessa ad orpello ingombrante da rimuovere ogni qual volta sia di ostacolo, non al riconoscimento pieno di un diritto bensì al soddisfacimento di un interesse. Sappiamo benissimo che tanti sono gli uomini probi chiamati in quest'Aula a svolgere l'importante e delicata funzione di legiferare: ci si vuole costringere a rinunziare a tale altissima funzione; ne esce umiliato il Parlamento e ferita la Costituzione. voi tanti uomini probi, accetterete di piegarvi all'interesse di un singolo? Qual è il limite della vostra sopportazione? Quando si riuscirà a recuperare la probità che vi appartiene? Oggi si è approvata una legge temporanea, in attesa dell'entrata in vigore di una legge costituzionale che ancora non esiste. Oggi, quindi, si è fatto ciò che non poteva essere fatto e chi l'ha chiesto ne è talmente consapevole da scrivere nella stessa legge che ciò è fatto per 18 mesi, perché poi la medesima materia dovrà essere regolata da una legge costituzionale. Sicché noi, investiti dalla Costituzione della nostra funzione, rinneghiamo per 18 mesi i principi costituzionali e mettiamo in quarantena la Costituzione: con una legge ordinaria abbiamo rinviato ad una costituzionale, ossia sovraordinata, che non esiste e non possiamo sapere né se o quando verrà approvata, né come sarà concepita e articolata. Gli uomini probi non possono non avvertire la gravità dell'insulto normativo e costituzionale compiuto: spero quindi che riflettano e si rendano conto che è stata ferita non solo la nostra funzione costituzionale di legislatori, ma anche la nostra dignità di cittadini uguali dinanzi alla legge; né la forza dei numeri potrà santificare il disprezzo della legge. *(Applausi dal Gruppo IdV).* Dobbiamo invero purtroppo constatare che massicce dosi di veleno sono ormai state instillate nel tessuto del quotidiano vivere degli italiani, essendosi altresì diffusi gli effetti del rancoroso e pericoloso crepuscolo di Silvio Berlusconi. Questo è un momento che tanto, forse più di noi suoi avversari, potrebbero fare gli uomini probi che non gli sono ostili. Agli uomini probi, non attaccati dal tarlo della corruzione delle coscienze, noi guardiamo con rispetto; non bisogna però troppo attardarsi nell'indulgenza: i cittadini sono stanchi della violenza delle parole e dei fatti. Vorremmo ritrovare la difficile serenità nell'affrontare, senza odiose contrapposizioni, i problemi del Paese e dei più sfortunati dei nostri concittadini. Ai tanti problemi se ne aggiunge uno ulteriore molto pesante: la crisi della democrazia, con la crescita di insane oligarchie, terreno fertile per l'autoritarismo. Vorremmo poterci liberare dalla infezione della mala politica, delle squalificate cortigianerie, degli approfittatori furbi di regime, dei nati servi. Vorremmo poter tornare ad essere un Paese normale, senza che tutto debba per forza essere eccessivo, e ritrovare la capacità, l'ingegno e la tenacia che hanno fatto grande e nobile un'Italia al contempo inadeguata. Compete a voi, uomini probi, ascoltare le vostre coscienze senza sottrarvi al dovere morale di assumervi le responsabilità dinanzi al Paese, perché noi non siamo un Paese normale. Il Presidente del Consiglio è orgoglioso del suo massimo esponente in Campania, lo tiene stretto come Sottosegretario all'economia e presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica; la stessa persona su cui pende un mandato di cattura confermato dal tribunale del riesame e dalla cassazione per collusione mafiosa con il sanguinario *clan* dei Casalesi. La magistratura arresta i mafiosi, il Governo se ne intesta il merito e il presidente Berlusconi li coccola, li protegge, se li prende in casa, da Mangano in avanti! Giaretta).* Bel messaggio agli onesti e alle forze dell'ordine, al senso del dovere dei tanti servitori dello Stato! Vi sembra normale ciò? Il Consiglio dei ministri, mortificando uno stordito ministro Maroni, non ha sciolto per infiltrazione mafiosa il Comune di Fondi e oggi 14 esponenti politici che non potevano essere candidati sono invece presenti nelle liste del PdL e collegate. Vi sembra normale ciò? Il Presidente del Consiglio ha una parossistica ossessione per la giustizia, ma se non fosse stato per le leggi *ad personam* sarebbe oggi un condannato a vari anni di carcere. È un Paese normale questo? Il Presidente del Consiglio ha affermato che il primo male dell'Italia sono i giudici - ora anche quelli del TAR - non la criminalità organizzata, non la corruzione, non la disperazione dei disoccupati e dei precari, non l'evasione fiscale, non lo sfascio idrogeologico e ambientale, non la crisi economica devastante per tantissime famiglie e imprese. No, il primo male dell'Italia sono i giudici. *(Applausi del senatore Applauditevi, siete complici! che voi condividete, per la sua protezione ai malfattori, per difendere se stesso da infamanti accuse, quale quella di aver costituito fondi neri per centinaia di milioni di euro e di aver corrotto un testimone. È un Paese normale questo? Berlusconi ha voluto la fiducia e sappiamo alcune cose che ancora farà: indebolire lo strumento delle intercettazioni telefoniche così da proteggere i malfattori, modificare alcune mirate norme del codice di procedura penale per limitare le indagini e le acquisizioni delle prove nei processi, far scarcerare alcune migliaia di imputati di gravissimi reati con la legge, alla quale non rinunzia, sul cosiddetto processo breve, ossia per decretare la morte di 100.000 processi. No, non è un Paese normale il nostro! L'Italia ha bisogno di governanti onesti, rispettosi della legge, determinati e convinti nella lotta al crimine, insospettabili, rispettosi dei diritti, accorti e attenti ai bisogni dei più deboli e sfortunati: tutto ciò che non è Berlusconi. L'Italia dei Valori crede nei valori sani - senatori Boscetto e D'Alia - e dice no all'arroganza, alla prepotenza, alla disonestà,

...agli uomini e alle donne dovrebbero stare a cuore questi valori e principi. Li tutelino con il loro voto. Fermino questa oscura e pericolosa deriva; fermino la rancorosa prepotenza di chi non ha alcun senso dello Stato, delle leggi e delle istituzioni.

che faticano, lavorano e producono nel rispetto dell'onestà e delle leggi!

e che non voglio ripetere per non urtare la sensibilità dei signori del centrosinistra. Consentitemi però di dire che questa è l'occasione, o meglio è una delle occasioni, per esprimere la posizione della Lega Nord in questa congiuntura politica nella quale, in tutta franchezza, ci pare che i problemi del Paese, quelli che stanno a cuore al nostro movimento in particolare, non siano alla nostra attenzione quotidiana come dovrebbero essere. essere. Il dibattito politico, infatti, si è incentrato nelle sedi istituzionali, sui giornali e sui programmi televisivi, solo su scontri politici, in molti casi strumentali, per garantirsi più visibilità in campagna elettorale. È stato detto e ripetuto dalla senatrice Finocchiaro che questo Paese sta marcendo. Noi non lo crediamo; noi non vogliamo credere a questo.

È per questo che, a maggior ragione, noi della Lega Nord siamo impegnati in mezzo alla gente, a partire dai nostri sindaci, per dare risposte concrete ai problemi reali della gente. Un esempio del clima infuocato da campagna elettorale che toglie l'attenzione dai problemi fondamentali è la questione delle liste. Al di là del merito specifico, hanno impegnato tutti noi, dirigenti di partito, in una azione convulsa e frenetica e ciascuno si è trasformato in un giurista o avvocaticchio di parte. La Lega Nord non si è certo appassionata alla vicenda, ma, se dobbiamo esprimere un'opinione che vada oltre i ricorsi al Tar, al Consiglio di Stato, alla Corte d'appello, mi sembra doveroso affermare come il nocciolo della questione fosse l'incongruità, la sproporzione, tra gli errori eventualmente commessi e la troppo severa punizione, che sottraeva il diritto di voto a milioni di cittadini estranei ai pasticci che si sono consumati. Del resto, è lo spirito con il quale si è mosso il Capo dello Stato, pensiamo tutti noi. A noi preoccupa questa deriva leguleica e cavillosa della politica ed anche dell'attività del Parlamento. È con questo spirito, con l'orgoglio e la voglia di tornare ad occuparci a tempo pieno di riforme, di federalismo, di occupazione, di sviluppo del Paese, di infrastrutture, di sicurezza, che ci accingiamo oggi a votare il provvedimento sul legittimo impedimento, gonfiato oltre misura dal clima elettorale. Altrimenti non mi spiegherei gli oltre 1.600 emendamenti presentati ad una normativa composta da pochi articoli; e non mi spiegherei le dichiarazioni di ostruzionismo rese dai Capigruppo di minoranza di Camera e Senato. Le sorti del Paese non possono certo dipendere da una questione procedurale, verso la quale non valgono le scontate invocazioni e i richiami costituzionali alla giustizia uguale per tutti. Nessuno qui vuole sfuggire alla giustizia, ma solo contemperare oggettive e diverse esigenze. Sul voto di fiducia, cari colleghi, devo dire che è diventato necessario anche se va sempre auspicato il dibattito parlamentare, perché è sin troppo palese e dichiarata la volontà ostruzionistica delle opposizioni. Provvedimenti importanti attendono quest'Aula già dalla prossima settimana, senza contare il freno che arriverà per gli impegni della campagna elettorale. Dobbiamo esaminare provvedimenti importantissimi come quello sugli enti locali, in scadenza, e quello sul sequestro dei beni dei mafiosi. Si auspica che questo ramo del Parlamento nella sua interezza sappia stabilire la gerarchia dei valori e le urgenze e tornare quindi ad occuparsi dei problemi che affliggono i nostri concittadini al di là di ogni appartenenza politica. E tra le risposte che vanno date c'è anche quella di garantire che il Presidente del Consiglio possa operare con assiduità e serenità, condizione primaria perché il Governo del Paese sia operativo e non intralciato dall'incompatibilità del calendario. In conclusione, il *latinorum* di Don Abbondio, Pippi calzelunghe, Alice nel paese delle meraviglie, ci interessano relativamente; sono favole: come le tante parole dette ieri ed oggi dal centrosinistra. A noi interessa lavorare sodo per riformare questo Paese, per premiare chi produce, chi lavora, e far cambiare la testa a chi vuole lasciare le cose come stanno. Il voto della Lega Nord Padania sarà,

le ragioni per cui, con assoluta convinzione e determinazione, voteremo contro la fiducia al Governo e contro questo assurdo provvedimento. Da voi ci aspettavamo di tutto, ma che sareste arrivati sino al punto di chiedere la fiducia su un atto che voi stessi sapete essere incostituzionale, tanto che la durata del suo contenuto è è pari al tempo necessario per il pronunciamento della Corte costituzionale; un atto la cui urgenza è dettata non da un bisogno del Paese, ma dal calendario delle udienze di ben precisi processi penali; un atto che non ha precedenti nella nostra vita parlamentare, tant'è che nessuno esponente di Governo ci ha spiegato perché sia stata posta la questione di fiducia; che sareste arrivati fino a questo punto proprio non l'avremmo immaginato. Sta accadendo qualcosa di una inaudita gravità. Lo abbiamo spiegato in questo dibattito, con gli interventi di tanti autorevoli colleghi. Sino ad oggi, se un uomo di Governo doveva presentarsi al giudice, ma dimostrava di avere un impegno legato alla propria funzione, documentandolo poteva ottenere un rinvio per il tempo strettamente necessario. Da oggi non sarà più così: il Presidente del Consiglio o un Ministro potranno decidere a proprio piacimento di sottrarsi a qualunque giudizio per un tempo lungo sino a 18 mesi, senza dover dimostrare nulla, senza che il giudice possa valutare, in barba al più elementare principio costituzionale per cui siamo tutti uguali di fronte alla legge. Altro che legittimo impedimento: questo è un illegittimo aggiramento della norma, care colleghe e cari colleghi! Un modo francamente spudorato per far rientrare dalla finestra, con legge ordinaria, quella impunità che la Corte costituzionale aveva fatto uscire dalla porta dichiarando incostituzionale il lodo Alfano. L'ennesima prova di una maggioranza e di un Governo che agiscono sempre e soltanto per difendere i propri privilegi. Le istituzioni, il Parlamento, il Governo per voi non devono servire il Paese; in questo momento, anzi, come noi crediamo, dovrebbero servire innanzitutto la parte più debole, più indifesa di questo Paese; no: per voi le istituzioni devono servire il sovrano. Vedete, è come se il Paese non esistesse. Vorrei farvi notare, cari colleghi, che dal 1° gennaio di quest'anno ad oggi questa ha dedicato 13 sedute e 46 ore prima per il processo breve, ora per l'illegittimo aggiramento, per risolvere uno ed un unico problema, sempre lo stesso, e non ha dedicato un minuto a chi sta perdendo oggi il posto di lavoro, un minuto a chi il posto di lavoro non lo trova, a chi non sa come mandare avanti la propria azienda! Oddio, è vero che quando vi siete occupati di lavoro, come è avvenuto la scorsa settimana, in quest'Aula,

dove si va a finire seguendo questa strada? E smettetela, smettiamola di raccontare la favola che state riformando la giustizia. Dio solo sa quanto bisogno c'è in questo Paese di riformare la giustizia, di renderla più rapida, più efficiente ed io dico anche più giusta, ma tutto quello che state facendo non ha nulla a che vedere con la giustizia al servizio del cittadino. State andando nella strada esattamente opposta: con una mano, il Governo fa balenare ai cittadini italiani il miraggio del processo breve, con l'altra mano allunga i tempi del processo che riguarda il Presidente del Consiglio, e l'unico risultato che produrrà questa altalena tra il falso processo breve e l'illegittimo aggiramento è che i processi riguardanti i comuni cittadini resteranno tali e quali, cioè insopportabilmente lunghi, mentre i processi di alcuni potenti saranno rinviati alle calende greche. Pagheremo l'impunità del Governo con la moneta sonante e costosissima di una giustizia ancora più lenta ed ancora più inefficiente; una giustizia, quella che piace a voi, come la descrisse Solone molti secoli fa: una una tela di ragno che trattiene gli insetti piccoli, mentre i grandi la trafiggono e restano liberi. Questa giustizia non ci piace! Certo, ci stiamo rendendo sempre più conto che questo modo di agire così arrogante ed ingiusto è ormai la cifra di questa maggioranza, e traspare ormai non solo negli atti, ma anche nei comportamenti politici. Penso al pasticcio di questi giorni sulle liste per le elezioni regionali. La prima cosa che, per la verità, tutti ci siamo chiesti è stata: come è possibile che a governare un grande Paese come l'Italia ci sia una forza politica che non sa neanche presentare le liste alle elezioni regionali? Ma poi si blocca un Paese, si sequestra il dibattito pubblico e si convoca d'urgenza il Consiglio dei ministri, quasi di notte, perché il partito del Presidente del Consiglio nel Lazio e in Lombardia ha presentato le liste senza rispettare le regole. Dunque, occorre fare un provvedimento, che peraltro si è rivelato inutile, per poterle riammettere abusivamente. Ma in che Paese siamo? Ma chi glielo spiega a quel giovane escluso da un concorso pubblico perché è arrivato un minuto dopo la scadenza? Chi glielo spiega a quella impresa esclusa dalla gara d'appalto perché manca un timbro? Chi glielo spiega che in questo Paese c'è chi le regole le deve rispettare e chi invece non ha questo problema, perché le può cambiare come e quando vuole, a proprio uso e consumo? Non illudetevi di poter utilizzare come scudo il Presidente della Repubblica. È noto a tutti che non è nelle disponibilità del Presidente della Repubblica il contenuto dei decreti che adotta un Governo. Al Presidente della Repubblica spetta il ruolo di garante delle nostre istituzioni, di interprete dell'unità degli italiani, di custode dei valori democratici. Il presidente Napolitano ha operato e opera sempre nel rispetto di questi principi ed anche in questa occasione ha agito con grande correttezza e grande responsabilità di fronte a un atto irresponsabile del Governo; non è caduto in nessuna trappola in buona fede. Cogliamo questa occasione per esprimere al presidente Napolitano tutta la nostra vicinanza e tutto il nostro apprezzamento, e lo facciamo oggi

quello della convenienza, del chi non è con me è contro di me, di chi crede che una maggioranza elettorale può legittimare e fare qualsiasi cosa. Questa è l'idea di democrazia che avete voi. Noi ne abbiamo un'altra: noi abbiamo l'idea di una democrazia che ha consentito al nostro Paese di crescere, di emanciparsi ed unirsi, persino nei momenti più drammatici, attorno a questa Costituzione. *(I senatori non è solo un complesso di regole, ma è il riconoscersi in una storia divenuta comune.

Signor Presidente, le chiedo di richiamare l'Aula a un atto di rispetto nei confronti della Costituzione. PRESIDENTE. Tutti abbiamo rispetto per la Costituzione, ci mancherebbe senatore. Dietro questa Costituzione, come diceva Calamandrei, si sentono voci lontane, si sentono voci di tanti grandi protagonisti, ma anche umili voci di lotta e di speranza di quanti hanno dato anche la vita per restituirci la democrazia. In nome di quei valori noi oggi difendiamo lo Stato di diritto contro questo Governo e contro questo ignobile provvedimento.

onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, sosteniamo questo provvedimento con convinzione e ci assumiamo tutta intera la responsabilità di approvarlo. Riteniamo che la legittimità dell'attività istituzionale di un membro del Governo, quindi di un organo di altissima rilevanza costituzionale, non debba essere lasciata alla libera interpretazione del giudice creando un inammissibile squilibrio e affidando ad organi esterni al Governo le decisioni sull'agenda dell'attività dell'Esecutivo. di legge - sia chiaro - non cancella i giudizi, perché durante l'intera durata del rinvio del procedimento la prescrizione rimane sospesa, in conformità con le norme del codice penale. Questa legge è una normativa ponte che guarda ad una riforma costituzionale che possa regolare i rapporti tra la politica e la magistratura. Non vogliamo garantire, né con questo né con altri provvedimenti che si discuteranno, immunità assolute; vogliamo, come in altri Paesi, regolare questi aspetti,

Per quanto riguarda le proposte di rango costituzionale che discuteremo, ce ne sono molte ed alcune forse dovranno aggiungersi al dibattito, ricordo, fra le tante qui al Senato, quella Chiaromonte-Compagna che, per i parlamentari, affida alla Camera di appartenenza l'eventuale decisione di sospendere un procedimento per la durata del mandato, per poi celebrare il processo al termine dell'incarico parlamentare. Si tratta di una proposta che non ha la paternità del nostro Gruppo, ma è tra le tante che meritano attenzione e rispetto. Puntiamo ad un equo contemperamento degli interessi in campo: la legittima azione del Governo, da un lato, e il corso della giustizia, dall'altro. Non vogliamo privilegi, non vogliamo immunità, ma delle norme che garantiscano una normalità di rapporti tra politica e magistratura. Avevamo ascoltato nei mesi passati, anche dai banchi del Partito Democratico, dell'UDC e perfino da alcuni settori della magistratura, considerazioni ben più serene di quelle di questi giorni. Ci auguriamo che su questi temi si torni ad atteggiamenti più riflessivi che possano lasciare il campo ad un confronto più maturo. Riteniamo queste norme pienamente conformi alla Costituzione e proseguiremo su questo tema in un confronto parlamentare. Il presente disegno di legge giunge dopo casi clamorosi, cari colleghi, che sono stati ricordati in Aula in questi giorni: fissazioni di udienze a raffica per il Presidente del Consiglio, persino nel giorno di chiusura della campagna elettorale,

Non ci nascondiamo dietro un dito e denunciamo questi fatti, così come li abbiamo denunciati nel passato, cari colleghi, quando anche Di Pietro - erano altri tempi!

ribadire in quest'Aula che contro Silvio Berlusconi si è abbattuta un'autentica persecuzione giudiziaria sin dalla sua discesa in politica

della sinistra che D'Alema e Di Pietro si sono serviti delle immunità europee per sfuggire a vicende che li hanno riguardati! *(Applausi

vedere come finirà il contenzioso sulla presentazione delle liste; cinque anni fa, all'ora giusta, avete presentato nel Lazio il candidato sbagliato: Marrazzo. Vergognatevi dello sfacelo nel quale avete fatto precipitare questa istituzione: l'ora era giusta, ma l'uomo era sbagliato!

Noi rispondiamo che siamo il primo partito d'Italia, che le elezioni regionali lo confermeranno e che nel Partito Democratico la crisi politica dei cattolici e di molti altri è ormai sotto gli occhi di tutti: è una considerazione politica che ho il diritto di fare in quest'Aula, nei confronti di chiunque e senza intimidazioni da parte di alcuno! Qualcun altro ha detto che noi non avremmo il senso dello Stato e che distruggeremmo le istituzioni. Abbiamo invece dimostrato il contrario affrontando tante emergenze: dalla ricostruzione dell'Abruzzo ai rifiuti di cui la sinistra ha ricoperto la Campania.

dai banchi dell'opposizione).* Voglio anche ringraziare la Presidenza per un atteggiamento di assoluta imparzialità e respingiamo le critiche che sono state rivolte con astio al presidente Schifani, che ha condotto con saggezza ed equilibrio questo delicato dibattito. e LNP).* Due ultime brevi considerazioni: qualcuno ha detto che questo provvedimento non era nel programma di Governo! contrastare l'uso politico della giustizia e garantire il corso serio ed equilibrato della giustizia è qualcosa di cui abbiamo sempre parlato. Non so se questo provvedimento fosse nel testo del programma, ma non era nemmeno nel vostro programma

In relazione all'andamento dei lavori, comunico che lo svolgimento del sindacato ispettivo, già previsto dal calendario per domani pomeriggio alle ore 16, è anticipato alla seduta antimeridiana di domani, alle ore 9,30. In relazione all'andamento dei lavori, comunico che lo svolgimento del sindacato ispettivo, già previsto dal calendario per domani pomeriggio alle ore 16, è anticipato alla seduta antimeridiana di domani, alle ore 9,30. Le Commissioni potranno convocarsi